Regolamento (ore 10). Seguito della discussione dei disegni di legge: (2287) Disciplina del cinema, dell’audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

Ieri non sono voluto intervenire sulle parole dell’ex presidente Napolitano, perché - come dicono giustamente alcuni colleghi di maggioranza - l’ex presidente Napolitano è intoccabile e di conseguenza non bisogna commentare le parole di un collega.

e tra le persone che fanno parte di questo Senato siano fondamentali. Penso che il rispetto, in quest’Aula e fuori, sia doveroso: rispetto, soprattutto, per il lavoro che viene svolto. Il Gruppo della Lega molto spesso non ha condiviso e non condivide le decisioni e il lavoro che viene portato avanti dai colleghi del Partito Democratico, ma ha sempre rispettato la dizione: “il lavoro che viene svolto nelle Aule parlamentari”. che, in modo anomalo, gira l’Italia a spese nostre per portare avanti le sue teorie referendarie. Questo signore ieri era a Treviso e, nella foga (un po’ anche nel nervosismo, visto e considerato come stanno andando le cose), ha fatto un’affermazione che ritengo indegna e brutta, non tanto nei confronti del senatore Centinaio, che conta come il due di picche,

perché al Nord gridano «Roma ladrona» e quando vengono qui stanno bene, perché la sera vanno a fare i festini e vanno a divertirsi”. Signor Presidente,

Caro presidente Zanda, penso che, nonostante le differenze di vedute, tra noi e voi vi sia sempre stata una parola che si chiama «rispetto»: noi mai e poi mai, in nessun momento, neanche con i militanti, siamo andati a denigrare il il lavoro che viene fatto dai colleghi del Partito Democratico. Abbiamo spesso detto che non eravamo d’accordo e che in Aula avremmo fatto le barricate: ma dire che c’è gente che viene a Roma a fare i festini e a divertirsi penso sia di uno squallore che la metà sarebbe già abbastanza.

Il signorino ha detto che non bisogna personalizzare il dibattito sul referen_dum e lui lo sta facendo, ancora una volta, attaccando dodici senatori della_ Repubblica italiana, eletti dai cittadini italiani, contrariamente a lui, che non è stato eletto neanche dal vicino di casa. (Applausi Il signorino dice che dobbiamo tornare a lavorare. Noi, signor Presidente, tutti noi, se dovessimo andare via di qui, torneremmo a lavorare, perché noi un lavoro lo abbiamo, contrariamente a lui che non ha mai fatto niente in vita sua. qui stiamo passando il limite. Prima l’ex presidente Napolitano insulta questo ramo del Parlamento, noi siamo stati in silenzio per rispetto nei confronti del presidente Napolitano e anche perché a me hanno insegnato che le persone anziane bisogna rispettarle e, ogni tanto, quando dicono qualcosa di poco lucido, bisogna lascia

siamo al limite. Non si possono insultare le persone. Abbiamo un dovere morale, noi dodici senatori della Lega, nei confronti dei nostri elettori e delle nostre famiglie. Non posso pensare che le famiglie di dodici senatori della Lega pensino che siamo qui a fare i festini.

Presidente, le chiedo di tutelarci nei confronti di una persona che in questo momento ha insultato un Gruppo parlamentare eletto dai cittadini italiani. Adesso basta. Presidente, l’intervento del senatore Centinaio merita una risposta e l’avrà, ma in questo momento penso che si debba tener conto anche delle delle esortazioni che sono venute dai banchi del suo Gruppo parlamentare. Infatti, in questo momento il Senato è impegnato nell’approvazione di un provvedimento importante, per cui io chiedo che si prosegua con l’esame di tale provvedimento.

nel momento in cui i lavori dell’Aula ci consentiranno di

favorevole perché intende sostenere la produzione di opere cinematografiche che possono valorizzare la cultura dell’integrazione

l’aiuto alle persone che sono in condizioni di difficoltà storiche, politiche e sociali e che vengono nel nostro Paese. giusto aiutare l’integrazione anche attraverso la sensibilizzazione del popolo italiano e questo è un ruolo che il cinema può L’audiovisivo riesce, più di tanti convegni, a rendere comprensibile non solo la necessità, ma anche la bellezza e la ricchezza del saper vivere insieme,

il finanziamento pari a 5 milioni di euro per l’anno 2017, volto ad alimentare la sezione speciale per l’audiovisivo del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese,

quindi è ormai parte integrante della proposta di legge che stiamo per approvare, l’inserimento di misure specifiche per i piccoli Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti.

È stato accolto un ordine del giorno similare della collega Serra, quindi è evidente che si è espresso parere favorevole affinché nelle scuole venga considerato il potere, la potenzialità del cinema, inteso come realtà di produzione di audiovisivo ma anche di interpretazione e comprensione dell’audiovisivo. Il cinema è didatticamente utilissimo per i ragazzi, sia per avere una maggiore possibilità di conoscenza di varie tematiche (da quelle scientifiche, a quelle storiche a quelle sociali),

in esame prevede dunque un piano straordinario per diffondere la cultura cinematografica nelle scuole. Teniamo presente che l’educazione all’immagine è

sia prevista l’educazione all’immagine e all’audiovisivo e quindi che ci sia realmente la possibilità di creare un

durante le proiezioni dei film, sia sulle televisioni private sia su quelle dello Stato.

di trasformarlo in ordine del giorno e pregherei il Governo di accoglierlo, perché si tratta di un tema di cui abbiamo parlato in Commissione e su cui siamo tutti d’accordo.

Dunque, di buon grado il Governo è disponibile ad accogliere un ordine del giorno che riguardi questa materia, valutando l’opportunità di

Grazie,

Il taglio dei titoli di coda parziale o totale, adottato da alcune emittenti, nella maggior parte dei casi per ricavare spazi temporali da destinare all’invio di spot pubblicitari, si rivela un atto atto irrispettoso nei confronti degli operatori cinematografici, con riferimento a tutte le componenti professionali, volontarie, logistiche, in forma singola o associata, agli enti coinvolti pubblici o privati,

al rispetto del principio di integrità dell’opera filmica mediante la citazione del lavoro dei tecnici, dei professionisti, degli artigiani, dei creativi, delle maestranze, dei luoghi utilizzati, degli enti degli enti locali che hanno agevolato la realizzazione dell’opera filmica anche allo scopo di promuovere il turismo legato alla conoscenza dei siti ospitanti

del Governo è conforme In tal caso, il Governo valuterebbe volentieri l’opportunità di tener conto dei contenuti.

Signor Presidente, le chiedo la verifica del numero legale, perché non è stato richiesto l’appoggio per la votazione elettronica.

avevo sottolineato come, di fatto, avessimo tutti dato per scontato questo stralcio. Naturalmente così è, ma è importante che in questa fase del dibattimento ci rendiamo conto di cosa stiamo facendo.

un elemento di ulteriore riflessione con un corpus sicuramente da approfondire, anche se all’interno di tale articolo vi sono tutti gli elementi per poter sviluppare delle corrette deleghe

Si tratta di investire nuove risorse, ad esempio con il tax credit, di rimettere le mani sul Fondo unico per lo spettacolo e di creare nuove opportunità di internazionalizzazione. Lo faremo seguendo delle metodologie, con i decreti legislativi, che coinvolgeranno molto entrambi i rami del Parlamento e quindi, da questo punto di vista,

che indicava chiaramente la strada della graduale eliminazione dell’utilizzo degli animali negli spettacoli, in particolare nelle attività circensi. Ora, lo stralcio dell’articolo

presentata dalla Commissione. È approvata. Per effetto dell’approvazione della proposta di stralcio S34.1, riferita all’articolo 34, le disposizioni ivi contenute confluiranno in un autonomo disegno di legge

la volontà del Governo di confermare la natura di collegato per tutti i provvedimenti normativi che si renderanno necessari per il riordino e il riassetto della disciplina dello spettacolo, preso atto dello stralcio ora votato.

Chiedo che il Governo, prima di assumere posizioni su argomenti così delicati, passi a una fase successiva in cui il tema del rapporto uomini e animali venga approfondito con un minimo di ragionevolezza e di buonsenso.

intervengo in dichiarazio- ne di voto sull’articolo 35 per evidenziare alcuni passaggi di natura finanziaria che a me sembrano non coerenti con la nostra normativa. Ancorché la 5[a] Commissione abbia dato

del testo di iniziativa del Governo, laddove la Commissione ha apportato alcune significative modifiche alle percentuali del credito di imposta da mettere a disposizione degli operatori.

se vi sono apporti di denaro singolo. Quindi è evidente che quella copertura finanziaria, ossia la cifra al centesimo indicata nell’articolo 35, non è sufficiente a coprire le nuove disposizioni del testo uscito dalla Commissione.

vuole agevolare - come dice lo stesso parere della Commissione bilancio reso per questo provvedimento - ed evitare alcune incrostazioni che possono derivare da un testo elaborato da chi tecnico del bilancio non è. La Commissione bilancio, soprattutto sugli

proprio ad a- diuvandum, nel senso della correttezza del testo e dell’agibilità delle stesse previsioni. In considerazione di tali motivazioni,

Alle ore 16,30 di martedì sarà solennemente commemorata in Aula, alla presenza del Capo dello Stato, la figura del senatore a vita, Presidente emerito della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. Nella seduta pomeridiana delle ore 17, il Presidente renderà comunicazioni sul calendario dei lavori. La Conferenza dei Capigruppo sarà convocata nel corso della stessa giornata di martedì.

onorevoli colleghi, signor Mini- stro, signor Sottosegretario, mi piace esordire, in queste brevi dichiarazioni di voto, con un ricordo personale di Gianluigi Rondi, cui probabilmente questa legge può essere dedicata, non fosse altro che per il ruolo, che ha ricoperto, nell’essere critico ma anche fautore delle fortune cinematografiche italiane. Gian Luigi Rondi ha nutrito amore e passione per il cinema, per tutto il contesto. E l’aver voluto questa Assemblea associarsi al mio emendamento 29.200, poi trasformato nell’ordine del giorno G29.200, con la benevolenza della relatrice Di Giorgi e dello stimatissimo sottosegretario Cesaro, sottosegretario Cesaro, ha sicuramente assunto un ulteriore significato, nel senso che il cinema, nelle sue varie componenti, comprese quelle di natura intellettuale, creativa e immateriale,

l’aspetto fiscale degli investimenti nel cinema. Ritengo che il ricorso al credito d’imposta possa rappresentare un

destinare le loro risorse allo sviluppo del settore. Altresì importante è stato l’ordine del giorno G26.203, approvato quasi all’unanimità da questa Assemblea, in merito alle sale cinematografiche. Accrescerne il numero sull’intera superficie del nostro Paese significa consentire maggiore fruizione da parte del pubblico, ma anche un aiuto indiretto e diretto all’occupazione e allo sviluppo della filiera cinematografica. Con questi sentimenti e auspicando così come è stato ben ricordato dal senatore Bruni, che mi ha preceduto la settimana scorsa su questo argomento - che il tema venga ancor di più approfondito e migliorato nel passaggio alla Camera, annuncio il voto favorevole dei Conservatori e Riformisti su questo provvedimento.

Signora Presidente, al fin siam giunti. Dopo sei giornate di Aula e tanti mesi fermi in Commissione - e non certo a causa del bicameralismo perfetto o del Senato dei fannulloni - arriviamo al voto finale. Il Governo e la maggioranza non si sono smentiti nemmeno questa volta. Gli annunci e gli spot non sono mai all’altezza dei contenuti. Questo disegno di legge ha avuto un iter travagliato (lo abbiamo visto tutti); gli annunci roboanti del Ministro hanno avuto solo l’effetto di archiviare il lavoro che la Commissione aveva iniziato su una proposta di legge parlamentare a prima firma della relatrice. Dopo gli annunci il nulla: un testo che è stato dimenticato, al punto da svolgere la relazione in Aula a luglio (per poter fare l’annuncio a Venezia) e ora in tempo per l’annuncio al Festival di Roma, riportato in Aula solo per tappare i buchi dei problemi della maggioranza sulle prescrizioni e il processo penale. Questa è la considerazione che hanno questo Governo, il Ministro e la maggioranza della cultura. Conosco da anni la relatrice e capisco bene il suo imbarazzo: non solo non è il suo testo, ma quello che presenta è un riempitivo di Aula per niente efficace. La legge per un settore così importante e rappresentativo come il cinema dovrebbe soprattutto occuparsi di cinema; dovrebbe inoltre comprendere, sulla scia della storia passata e recente della nostra cinematografia, che qualità, creatività e innovazione sono il capitale culturale su cui investire. Il testo non disegna una prospettiva per il settore cinematografico: nel testo in discussione l’opera cinematografica diventa opera audiovisiva, e di conseguenza il risultato, che è il vero obiettivo del Governo, è sovvenzionare un po’ di più tutti i grandi interessi, dai produttori di videogame (che il linguaggio burocratico definisce “contenuti videoludici”) alle fiction tv, a favore dei grandi e potenti, e a danno dei piccoli, ancora una volta e come sempre. Siamo partiti dalla costituzione di un Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive, per far nascere nuovi cinema, modernizzare le sale già esistenti e soprattutto sostenere le nuove opere cinematografiche e audiovisive,

La percentuale attribuita alle eccellenze e ai prototipi scende notevolmente, essendo compresa nella quota una sequenza di voci che attengono alla promozione in Italia e all’estero. tra le righe le scelte del Governo: una generosa mano offerta ai produttori e alle loro associazioni, uno schiaffo all’universo degli autori e delle piccole strutture. Insomma, il rischio di premiare sempre i soliti diventa realtà. Si poteva, ad esempio, ad esempio, scegliere di tutelare le opere difficili, ma anche questo sembra impossibile in questo Paese. Sono state ridotte persino le risorse alle associazioni di cultura cinematografica non più finanziate con un contributo annuale per la loro attività

Non siamo stati tranquillizzati dalle parole della relatrice sul non avere accettato un emendamento sulla parità di genere, perché una cosa sono le buone intenzioni, altro le norme di legge. Si prevedono contributi per la ristrutturazione di sale e apertura di nuove sale, ma non si pongono rigidi vincoli urbanistici per evitare la la costruzione dei multisala o meglio dei centri commerciali con sale cinematografiche. Anzi, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - in virtù del voto del 4 dicembre, in questo disegno di legge si è aperta una grande trattativa possono introdurre comunque previsioni urbanistiche in deroga per le sale e i centri culturali multifunzionali. Insomma la legge non punta come dovrebbe sulla qualità, sulla creatività e sull’innovazione del cinema indipendente; una denuncia che ha fatto a luglio il direttore del Festival di Venezia Barbera, il quale, in piena conferenza stampa, ha parlato di riduzione della qualità media della produzione italiana, di cui i produttori sono consapevoli, ma - si sa - i soldi sono pochi e si finanzia senza scelta. Come è stato scritto da autorevoli e attenti commentatori del testo, di legge manca la parola “passione”, manca la capacità di suscitare passione per il futuro, nei ragazzi, negli spettatori e nel pubblico: tutto è concentrato sulla produzione e su pochi produttori. Il cinema vive se il pubblico è attento, coinvolto, se trasmette cultura, se è accessibile a tutti. Ad esempio, sarebbe prevedere misure fiscali per dimezzare i costi degli abbonamenti mensili alla sale cinematografiche, come avviene in Francia. Nessuna politica è stata prevista sui costi del biglietto. E non possono bastare le giornate del cinema a prezzi scontati, ma serve una politica diversa sui costi dei biglietti. biglietti. Oggi i dati ci dicono che i ragazzi non vanno a cinema come e quanto vorrebbero perché non possono permetterselo. 2016 Non tralasciamo poi il famoso articolo 31-bis che è stato introdotto: in nome della stabilizzazione del precariato in un settore che vive di precariato, abbiamo votato e introdotto il jobs act anche nel cinema. C’è poi il tema dell’alfabetizzazione audiovisiva, nel testo ridotta a “educazione all’immagine”, da insegnare genericamente a scuola, senza specificare come, dove e da chi. Ci è stato ampiamente illustrato ed è stato anche oggetto di una discussione questa mattina in Assemblea con i soliti richiami alla legge n. 107 del 2015. Non abbiamo tuttavia capito se sarà una materia vera e propria o una competenza trasversale. Inoltre - a nostro avviso - l’alfabetizzazione audiovisiva dovrebbe essere considerata un vero e proprio diritto di cittadinanza. Siamo dinanzi a un ennesimo disegno di legge delega con troppe deleghe, che avrà bisogno di decreti attutivi, che saranno preparati ancora una volta nel chiuso delle stanze del Ministero, come questo testo, senza alcun vero confronto pubblico per ascoltare le tante proposte e disegnare il futuro del cinema, piuttosto che fotografare il presente e la gestione degli ultimi anni. Questo provvedimento non migliora lo stato di salute del cinema italiano. Non basta dare un po’ di soldi in più e nemmeno tanti soldi in più, perché ricordiamo che la produzione di film italiani è diminuita, i registi sono quasi esclusivamente uomini e il mercato delle sale e della tv in Italia (anche nella rete pubblica e generalista) continua a essere dominato da produzioni americane. Da anni eravamo in attesa di una legge sul cinema ispirata al modello francese.

per dare una nuova normativa al settore del cinema, particolarmente importante e nel quale l’Italia ha una lunga tradizione, ma che sta soffrendo un momento difficoltà. Questo disegno di legge prevede interventi ad ampio spettro che definiscono i principi fondamentali dell’intervento pubblico a sostegno del cinema e dell’audiovisivo, in quanto settore idoneo a contribuire alla definizione dell’identità nazionale, alla crescita civile, culturale ed economica del Paese. un provvedimento che disciplina in maniera sistematica il settore cinematografico e della produzione audiovisiva, razionalizzando le misure di investimento attualmente previste; interventi che si rendono necessari

se volessimo utilizzare una metafora vicina al mondo del cinema, noi potremmo definire il testo di legge in esame un film già visto, con un copione trito e ritrito che si sussegue negli anni con stratificazioni normative che poi non trovano seguito nei decreti attuativi. E nel 2016 ci ritroviamo di fronte all’ennesimo tentativo di riordinare la normativa e riformare il comparto del cinema. Non vorrei deludere gli operatori del settore che si ritroveranno tra poco al Festival del cinema di Roma, perché questo disegno di legge rischia di naufragare per mancanza di tempi adeguati. Infatti, siamo solo al primo passaggio in Senato di un testo che dovrà essere trasmesso alla Camera

l’applicazione di qualsiasi norma nel testo è costantemente demandata, giustamente, ai decreti attuativi, il più importante dei quali, riferito all’articolo 11, comma 5, con cui si provvede al riparto del fondo per il cinema e l’audiovisivo, di nuova istituzione in questo disegno di legge, non prevede un termine di emanazione, come se il Governo sapesse già che forse il tutto è destinato a finire nel Mare dei Sargassi. Ma ripercorriamo un po’ le tappe del provvedimento in esame, che parte con un’iniziativa parlamentare della senatrice Di Giorgi e del senatore Giro, per poi

Franceschini è completamente sbilanciato sull’aspetto industriale. E, infatti, in esso sono preponderanti gli articoli che si occupano di tax credit, di misure finanziarie e di altre misure a sostegno del cinema. Certo, è necessario sostenere il cinema, anche se ci verrebbe da dire che poi sono necessari anche i decreti attuativi a sostegno del cinema. Nella legge di stabilità del 2016, che abbiamo esaminato a dicembre 2015, era prevista una modifica del tax credit con ri- ferimento agli investitori esterni al settore. Questi avrebbero beneficiato di un credito d’imposta pari al 40 per cento del capitale investito. I decreti attuativi, per rendere realizzabile questa norma, erano attesi per il 1° aprile 2016. ha inviato una lettera a tutti i membri della Commissione dicendo che i decreti attuativi non erano ancora stati emanati e non lo sono ancora oggi. La non emanazione dei decreti attuativi ha fatto sì che la direzione generale del cinema abbia sospeso in modo indiscriminato le procedure per i produttori cinematografici per l’accesso al tax credit esterno,

con un grave danno per i produttori che si trovano a corto di liquidità per la copertura dei costi iniziali di produzione delle opere cinematografiche. Quindi, di che cosa stiamo parlando?

ha detto che questa non è una delega, ma è chiaramente una riforma e che l’enorme lavoro fatto in Commissione ne é la prova. Collega, mi dispiace, ma non è così. Questa è una delega mascherata, perché in questo disegno di legge non si fa altro che rimandare a decreti ministeriali e a successivi a successivi decreti attuativi dove saranno decise delle cose importantissime. Quindi, se questo disegno di legge fosse stato tale e non fosse stato una delega prese delle decisioni fondamentali come, per esempio, la definizione dei parametri per l’erogazione dei contributi automatici. Su questo punto ci ritorno, perché uno di questi parametri, che è ben chiaro nel disegno di legge, è la bigliettazione. In Assemblea avete respinto

con dei criteri comparativi basati sul numero delle sale in cui il film è stato distribuito e sui giorni di presenza nelle sale, il parametro della bigliettazione finirà per premiare i soliti big e blockbuster, a discapito dei film

È stata prevista una norma per la distribuzione internazionale e non per la distribuzione nel suo complesso. Si tratta di una norma che prevede un rialzo della percentuale del tax credit per i produttori che sono anche di- stributori, ma si fa specifico riferimento alla distribuzione internazionale, mascherando un regalo con la necessità per il nostro comparto del cinema di internazionalizzarsi, di implementare e sviluppare le coproduzioni a livello internazionale. Perché si fa un regalo? Perché, guarda caso, gli operatori del cinema sanno benissimo che oggi la distribuzione internazionale è affidata a imprese di limitate dimensioni, ma ma è recente la nascita, la costituzione di una nuova società, la «True Colours», già ben strutturata - vi invito ad andare a vedere chi sono i componenti di questa «True Colours» - che evidentemente godrà di gran parte dei benefici legati alla distribuzione internazionale: un bel regalo ad altri big mascherati dietro un nuovo nome. sono i contributi selettivi: la relatrice era d’accordo nel mantenere la percentuale del 25 per cento per i contributi selettivi, ma queste percentuali sono state ribassate tra il 15 e il 18 per cento. Addirittura è previsto

in questo disegno di legge c’è anche una mancanza di trasparenza al Consiglio superiore per il cinema e l’audiovisivo. Non si sa come la rete nazionale delle cineteche potrà realizzarsi a costo zero; rischierà di dare linfa a un nuovo oligopolio distributivo, con la nascita di un nuova realtà distributiva, con Sky Italia, Indiana, Italian International film, Cattleya, Cattleya, Wildside e così via. Noi confidiamo che ci sia un passaggio alla Camera di questo testo. Confidiamo che esso possa trovare il suo naturale epilogo in un dibattito parlamentare che si sposterà alla Camera, nei confronti del quale - spero i relatori e il Governo saranno più propensi all’ascolto. Per questo, unicamente per questa ragione, il Movimento 5 Stelle esprimerà voto di astensione sul provvedimento al

Il difetto di questa maggioranza politica e di questo Governo lo conosciamo: il Parlamento non conta niente o conta ben poco. hanno l’ossessione di questo referendum per superare il cosiddetto bicameralismo paritario, inventandosi un bicameralismo imperfetto, perché il Senato non viene abolito, ma se fosse per loro con un tratto di penna abolirebbero sia la Camera che il Senato, tanto - come ci ha ricordato Centinaio (anzi, colgo l’occasione per esprimere la mia solidarietà al Gruppo della Lega) - siamo tutti degli sfaccendati. Quindi, l’elefante ha partorito un topolino, ma dato che sono cattolico praticante ho studiato buoni testi, fra cui quelli di San Tommaso e talvolta San Tommaso ci insegna che bisogna scegliere il male minore per non produrre un male peggiore. Quindi noi esprimeremo un voto favorevole, anche perché se uno si presenta da me

confermiamo, stabilizziamo, potenziamo, codifichiamo sei crediti d’imposta, sei tax credit per la distribuzione, per la produzione, per l’esercizio, per l’attrazione degli investimenti stranieri, per la diffusione del cinema italiano all’estero», è chiaro che io dico “sì”, “ci sto”, “sono d’accordo”. E voglio esprimere davanti a questa proposta un pegno di fedeltà. Mi sarei però aspettato una maggiore disponibilità della maggioranza e del Governo rispetto ad una serie di iniziative emendative per dare visione a questa legge. Tanti, tantissimi soldi, ma pochissima visione. Ha ragione la rappresentante di SEL: potevamo fare molto di più. Ma il nodo il nodo era il Centro nazionale per la cinematografia; era la proposta del PD di istituire il Centro nazionale del cinema e dell’audiovisivo, dando agli addetti ai lavori del cinema piena autonomia: lo fanno loro il cinema, si dessero loro le regole. Peraltro, il fondo dei 400 milioni viene alimentato con un prelievo dell’11 per cento dall’IRES e dall’IVA di tutti gli stakeholder, cioè degli addetti ai lavori:

6 Ottobre 2016 gestire in autonomia con il controllo del Parlamento, delle Commissioni di merito. Potevamo individuare dei passaggi di verifica e di controllo della qualità, perché dopo il disastro degli anni Novanta con il fondo di garanzia di Veltroni che dava soldi a tutti per film mai fatti, è chiaro che qualche criterio e qualche vincolo potevamo anche codificarlo. Ha ragione

il fondo dei 400 milioni annui viene gestito attraverso un decreto ministeriale che stabilirà i requisiti di ammissione e i casi di esclusione dal fondo. tutti i tax credit, come oggi (quindi non cambierà nulla), vengono gestiti da un decreto ministeriale. Dopodiché abbiamo le deleghe vere e proprie con i decreti legislativi, con i decreti legislativi, che verranno predisposti grazie al Ministro che dovrà promuoverli e proporli attraverso un decreto ministeriale. Quindi il decreto ministeriale è un totem che resta. E dovremo discutere sul registro cinematografico, sulla censura, sui broadca_ster; quindi è una delega in bianco._ Perché dunque Forza Italia vota a favore? Perché noi non possiamo fare un passo indietro: è meglio assicurare al cinema italiano queste risorse, che sono attese da lunghissimo tempo. Cercheremo di seguire tutto il processo successivo nella predisposizione dei decreti ministeriali, perché credo che il Ministro abbia l’interesse a coinvolgerci e sentire soprattutto gli operatori prima di predisporre tutti questi decreti ministeriali per i tax credit, per il fondo selettivo, per i contributi automatici. Credo che si possa fare un percorso insieme. Tornare indietro sarebbe stato deleterio per il cinema italiano in un momento di grande sofferenza, perché la bigliettazione è lì davanti a noi e i problemi ci sono.

un anno fa partecipò ad un convegno. È morto a gennaio, ma fino all’ultimo ha lavorato per il cinema. Non era un uomo di centro e neppure di destra. Anzi, ha avuto delle responsabilità nella sinistra essendo stato ministro per la cultura

da noi non c’è mai stata e temo che la stiamo ancora aspettando. Quindi, il suo giudizio sul disegno di legge in esame non sarebbe così positivo, però anche lui, in quell’occasione,

a un altro grande del cinema italiano, che non lo ha fatto ma ci ha insegnato a leggerlo e capirlo: Gian Luigi Rondi, un grande critico che

relatrice e il confronto con il Ministro e il Sottosegretario, che è stato spesso presente e ha seguito i nostri lavori, hanno portato a un buon testo. Credo di essere

come gli operatori non avrebbero sperato. Si tratta di un passo decisivo, molto forte e determinato del Governo, che ha messo sul tavolo fondi cospicui e la disponibilità ad affrontare un iter parlamentare produttivo e utile che andasse nell’interesse

per parlare di cinema nella scuola ed educare i ragazzi al cinema. Abbiamo inserito la possibilità della cessione del credito di imposta per aiutare i piccoli, quelli che magari hanno la qualità, ma non la capacità finanziaria, e lo abbiamo fatto inserendo strumenti alla portata di tutti. Abbiamo deciso di supportare le piccole sale cinematografiche; nei piccoli centri ci saranno molti «cinema Paradiso» nuovi, che riapriranno e che potranno essere fruiti da tanti italiani. Signor Ministro, consegnerò il testo scritto del mio intervento; mi auguro che lei abbia modo di leggerlo. Oggi dichiaro,

Signora Presidente, sono consapevole sia dell’ora che del giorno quindi prometto che sarò conciso. Credo, però, davvero di dover ringraziare tutti coloro che hanno collaborato al

hanno dimostrato che su alcuni terreni ci può essere uno sforzo comune. Il percorso è stato veramente costruttivo. Questo provvedimento è atteso da molti anni, da qualche decennio, dal mondo del cinema

in modo significativo, ma introduce nel nostro ordinamento un ancoraggio preciso. Tante volte è stato citato il modello francese, per cui i 400 milioni di cui parliamo in realtà potranno essere di più perché sono ancorati all’11 per cento di IRES e IVA che devono che devono versare le imprese che si occupano a vario titolo di contenuti, cioè i contenitori. Finisce la discrezionalità, quindi tutte le polemiche che hanno caratterizzato i Governi nei vari colori; i film di rilevante interesse culturale come strumento discrezionale per finanziare quel film e non quell’altro. Qui il contributo è tutto automatico, con i sei tax credit, ad eccezione di una quota importante che in valore assoluto è più di quanto viene destinato oggi (dal 15 al 18 per cento) per le opere prime, per i giovani autori. A tal proposito, rispondendo ad alcune richieste che sono state fatte, spero che nella legge di stabilità - ma non posso assumere un impegno: io mi impegno a provarci, poi la volontà è del Governo e del Parlamento complessivamente - alcune spese fisse dello Stato (mi riferisco al Centro sperimentale di cinematografia, all’Istituto Luce-Cinecittà, alla Biennale) possano trovare un finanziamento in un capitolo ad hoc, che di conseguenza faccia aumentare questa quota discrezionale di contributi selettivi. Poi ci sono le sale, gli interventi importanti per la scuola; scompare la censura. Insomma, mi pare veramente un grande passo in avanti e di questo ringrazio di cuore il Senato.

Presidente, credo non possa cadere nel vuoto l’intervento svolto dal capogruppo Centinaio ad inizio seduta. Successivamente, il Presidente del Gruppo Par- tito Democratico ha rinviato a un momento che non può che essere all’interno di questa seduta, altrimenti vorrebbe dire assecondare e dare ulteriore credito al dileggio tenuto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti dei senatori, legittimamente eletti, che rappresentano la Lega Nord e che si impegnano quotidianamente in maniera corretta corretta nel proprio mandato. Su questo riformulo la questione e chiedo al Presidente del Partito Democratico di assumere una posizione nella dignità anche dell’istituzione nella quale operiamo tutti.

che praticamente è la sublimazione di un vero e proprio grido di dolore per la morte del proprio figlio, il giovane Davide Gaetano D’Accolti, un brillante studente ucciso lo scorso 21 febbraio da un pirata della strada, risultato poi positivo sia all’alcol test che alla cocaina ed ai cannabinoidi e che percorreva contromano la statale n. 16 all’altezza di Torre a Mare, in provincia di Bari. I genitori del giovane Davide non si limitano a chiedere giustizia, ma si stanno impegnando in una nobile e meritoria opera di sensibilizzazione, affinché le istituzioni tutte di ogni ordine e grado operino con strumenti ed iniziative volte a ridurre il numero di incidenti, come quello tragico accaduto al proprio figlio. Chiedo quindi a lei, signora Presidente, di sollecitare il Ministro dell’interno a fornire una risposta a questa interrogazione. Lo chiedo anche per difendere la dignità di quei genitori che aspettano un segnale dal Parlamento.

Signora Presidente, nella grande caserma di Bagnoli di Sopra, in provincia da Padova, sono oggi ospitati - o sarebbe meglio dire ammassati - 850 richiedenti asilo. Giunge notizia che è in atto la ristrutturazione di un’altra palazzina, evidentemente per aumentare ancora il numero degli ospiti. Ogni volta che si ha notizia di nuovi sbarchi, i cittadini di Bagnoli di Sopra sanno che, in capo a pochi giorni, arriveranno nuovi migranti. Malgrado l’amministrazione comunale di Bagnoli di Sopra - un paese di tremila abitanti - abbia sempre cercato di collaborare al meglio con la prefettura, la situazione sta diventando insostenibile. Le pubbliche promesse del ministro Alfano di svuotare la caserma di Bagnoli di Sopra finora non hanno avuto alcun seguito. Lo stesso dicasi per la caserma di Cona, un altro piccolo Comune situato a pochi chilometri da Bagnoli di Sopra, dove vivono mille ospiti.

perché sono mortificanti per i richiedenti asilo, che in tali strutture non possono svolgere alcuna seria attività di integrazione, e perché suscitano grande inquietudine fra le popolazioni circostanti. Va invece potenziata l’accoglienza diffusa, che si sta dimostrando in grado di garantire seri percorsi di integrazione, coinvolgendo in modo più diretto i Comuni, il terzo settore, i privati cittadini. Inoltre, vanno drasticamente accorciati i lunghissimi iter burocratici per la concessione o il diniego dell’asilo: pur garantendo a ogni migrante il diritto di ricevere un giudizio equo, i tempi vanno limitati e le procedure snellite. È sbagliato, infine, un approccio assistenzialistico ai richiedenti asilo, che molti italiani in modesta condizione economica considerano come dei mantenuti, che godono di privilegi a loro negati. Per questi giovani andrebbero formulate ragionevoli proposte di lavoro, modificando a tal uopo l’attuale normativa. L’Italia, lasciata sola dall’Europa, sta facendo un lavoro fantastico, salvando la vita a migliaia di persone che cercano di attraversare il Mediterraneo: addirittura diecimila nei soli due giorni 4-5 ottobre. Non mortifichiamo questa grandiosa opera di salvataggio, gestendo male la fase successiva di valutazione e di integrazione. Dobbiamo voltare pagina, attuando politiche migratorie credibili agli occhi dei cittadini comuni, specialmente di quelli più poveri. Non lasciamo inoltre che i Comuni, specialmente quelli piccoli, siano lasciati soli a portare pesi obiettivamente insostenibili. Signora Presidente, a pochi giorni dalla dolorosa perdita del senatore Marco Conti, ci ha lasciati un’altra preziosa personalità della politica abruzzese. Si e spento infatti Corradino Di Stefano, già senatore della Repubblica, abruzzese, di Castelli. È scomparso ad ottantacinque anni nella sua casa, nel paese che tanto amava e di cui era stato sindaco dal 1964 al 1990 per cinque mandati. Prima consigliere comunale, poi sindaco, presidente della Comunità montana, componente degli organismi dirigenti della Democrazia Cristiana e poi senatore per tre mandati dal 1984 al 1992,

Amava la sua terra in una maniera genuina e direi viscerale. La sua Castelli, le ceramiche, i monumenti, le piccole economie locali erano argomento di azioni e battaglie politiche. Legatissimo alla sua terra, si adoperò in tante battaglie per il lavoro e lo sviluppo del Mezzogiorno. Il Museo delle ceramiche di Castelli,

seppur momentaneamente, dato un aiuto economico proprio per la situazione dei call center. perché il Partito Democratico non ha aderito a questo bando, lo ha fatto scadere e oggi si permette anche di spendere qualche parola. Manda cioè al macero le persone e poi

soluzione a questa incresciosa situazione che, in realtà, ha visto l’azienda non rispettare diversi patti. Non è possibile procedere ancora così, Presidente, perché queste aziende vengono in Italia, la possibilità di lavorare e guadagnare, ci offrono magari servizi, dopodiché vanno all’estero ad aprire altre aziende e continuano ad offrire servizi,

non pervenuta e non accettata da parte del presidente De Luca; ciò mi lascia veramente sconcertato. La seconda proposta è che si apra immediatamente questo tavolo al Ministero.

fermi questi incresciosi episodi, che vedono queste aziende venire in Italia a vendere i prodotti ad aziende statali italiane, avendo i lavoratori da tutt’altra parte.

eseguire un’ordinanza di custodia cautelare per quattro persone. Si trovava perciò lo scorso 27 di settembre a Mariano Comense e con i colleghi

di una casa. Sebastiano è risultato gravemente ferito al cervello. Due giorni dopo, il 29 settembre, è stato operato all’ospedale Sant’Anna di Como. La prognosi Grazie Nord, voglio fare gli auguri di pronta guarigione all’agente Sebastiano Pettinato, esprimere sentimenti di vicinanza alla moglie, con la quale si è da poco sposato, nonché di solidarietà ai colleghi di Sebastiano che lavorano presso la questura di Lecco e a tutte le Forze dell’ordine che lavorano in Italia e vedono, purtroppo, aumentati i propri rischi professionali. Il marocchino sta cercando, attraverso il suo legale (uno di quelli che si occupa di queste situazioni e della malavita), di alleggerire la sua posizione,

ma in abiti civili. Voglio fare una volta per tutte un appello al Governo, al Ministro dell’interno e al Ministro della giustizia affinché i rischi professionali degli agenti delle Forze dell’ordine tendano a diminuire e i rischi per i delinquenti che vogliono, appunto, delinquere, possano aumentare: una volta arrestati, devono finire nelle patrie galere e lì scontare

a centinaia di migliaia, che operano nel nostro Paese per difendere i cittadini e che in questa occasione sono stati purtroppo colpiti. Penso di interpretare il pensiero di tutta l’Assemblea, e non solo del Gruppo della Lega Nord, nel ribadire i sentiti auguri di pronta guarigione a Sebastiano Pettinato, a che possa tornare quanto prima possibile a lavorare con i suoi colleghi per difendere la sicurezza di tutti cittadini italiani. (Ap- plausi dei rivolge sicuramente gli auguri di pronta guarigione a questo agente. Siamo ovviamente vicini alla moglie e alla famiglia e sappiamo che, sull’altro versante, la magistratura farà il suo lavoro, puntualmente come sempre.

parlano queste interrogazioni? Parlano della sicurezza, non di tutti i cittadini italiani, ma di due milioni di cittadini italiani, che sono affetti da epatite C e che non si possono curare,

familiari, nel senso che dalla Consip c’è stato il trasferimento all’Aifa di uno che faceva le gare per l’Aifa e il suo trasferimento è stato preceduto dall’assunzione della moglie e di molti collaboratori del Ministero della salute, Grazie

si guarisce. Tutti i giorni ci sono centinaia di persone che muoiono di epatite C e noi dobbiamo curarli, con un farmaco che in altri Paesi costa 800 euro e da noi

Grazie